La Presidenza ha appena ricevuto una comunicazione con la quale uno dei due relatori, il senatore Mazzatorta, informa di non poter essere presente in Aula per ragioni di salute. Il senatore Mazzatorta aggiunge che è sua intenzione rimanere relatore del disegno di legge in questione, in caso di auspicabile rinvio, considerato il suo interesse per la materia e la disciplina che lo regola. La Presidenza ritiene che la richiesta del senatore Mazzatorta debba essere accolta, come gesto di cortesia nei confronti del relatore. La discussione del provvedimento è pertanto rinviata ad altra data, che verrà indicata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

sarò relatore soprattutto per gli aspetti che interessano la 3a Commissione e, da questo punto di vista,

conseguente all'inquinamento marino causato da residui di carburante utilizzato per la propulsione delle navi. Come si può rilevare dall'oggetto, sotto alcuni profili è di più precipua competenza dei colleghi dell'8a Commissione.

il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, intende autorizzare l'adesione dell'Italia alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, fatta a Londra nel marzo del 2001 ed entrata in vigore a livello internazionale nel novembre del 2008, con il coinvolgimento di 44 Stati, che rappresentano circa il 78 per cento del tonnellaggio navale mondiale. Tale Convenzione, negoziata in seno all'Organizzazione marittima internazionale, intende colmare un vuoto della disciplina internazionale nella lotta contro il fenomeno dell'inquinamento marino provocato dal trasporto marittimo, prendendo in considerazione, in particolare, l'inquinamento provocato dalla fuoriuscita e dal versamento in mare di petrolio utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi. Essa è stata pertanto adottata per assicurare alle persone danneggiate dalla perdita di carburanti utilizzati dalle navi un risarcimento congruo, adeguato e tempestivo; contiene inoltre misure di salvaguardia volte a prevenire e a limitare tali danni. Complessivamente la Convenzione si compone di un preambolo e di 19 articoli; il suo campo di applicazione comprende i danni occorsi nel mare territoriale e nelle zone economiche esclusive - o in aree marine equivalenti - di pertinenza degli Stati aderenti, mentre non riguarda i danni causati da inquinamento da idrocarburi - che formano l'oggetto della Convenzione di Londra del 1969 - né quelli subiti da navi da guerra o che appartengano ad uno Stato e siano utilizzate esclusivamente per un servizio pubblico non commerciale. La Convenzione sancisce il principio della responsabilità oggettiva dell'armatore della nave per i danni causati dall'inquinamento, a meno che egli non fornisca le prove che il danno sia stato causato da atti di guerra o da ostilità, da fenomeni naturali di portata eccezionale, da azioni o omissioni intenzionali di terzi soggetti - comprese le persone che hanno subito i danni - o da negligenze di pubbliche autorità responsabili di aiuti alla navigazione. Il fulcro della disciplina dettata dalla Convenzione è contenuto nell'articolo 7, che - ricalcando quanto stabilito nella già citata Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile conseguente a inquinamento provocato da petroliere - prevede l'obbligo per il proprietario delle navi di stazza superiore a 1.000 tonnellate di sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria per un importo pari a quello del limite di responsabilità applicabile e, comunque, non eccedente l'importo fissato dalla Convenzione del 1976 sulla limitazione di responsabilità per crediti marittimi. Il certificato di attestazione della validità dell'assicurazione, che la nave deve conservare a bordo, è rilasciato dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave o, nel caso di navi registrate in Stati terzi, dall'autorità di uno qualsiasi degli Stati aderenti alla Convenzione. Tali Stati, peraltro, si impegnano a non rilasciare l'autorizzazione al commercio alle navi battenti la propria bandiera, sottoposte agli obblighi stabiliti dalla Convenzione, che non siano munite di certificato di assicurazione; essi sono tenuti altresì a vigilare che ogni nave in entrata o in uscita da uno dei loro porti, che rientri nei requisiti fissati dalla Convenzione, sia in possesso di un'assicurazione o di una garanzia corrispondente, a prescindere dal suo Stato di immatricolazione. Un'altra norma di particolare rilievo, contenuta nella Convenzione, è quella che introduce la possibilità di presentare la richiesta di risarcimento dei danni da inquinamento direttamente all'assicuratore, il quale può avvalersi dei mezzi di difesa spettanti al proprietario, ivi incluso il diritto di limitazione di responsabilità come regolato nell'Accordo. Ulteriori disposizioni riguardano, tra l'altro, gli avvenimenti che coinvolgono più navi, la competenza giurisdizionale, le clausole di prevalenza, le procedure di sottoscrizione, ratifica ed entrata in vigore dell'Accordo. Quanto al disegno di legge di ratifica, segnalo come l'articolo 3 individui nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorità responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione, mentre in base all'articolo 4 è attribuita al Ministro dello sviluppo economico la competenza a individuare l'ente abilitato al rilascio del certificato assicurativo dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a disciplinare, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di richiesta e di rilascio del certificato e il relativo costo. l'articolo 5 vengono introdotte norme volte a coordinare il decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, relativo all'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con la disciplina ora introdotta. Si segnalano in particolare, le modifiche relative agli articoli 1, 6 e 12 di tale decreto, finalizzate, rispettivamente, ad adeguare le definizioni, ad aggiornare le norme sul certificato assicurativo e a ridefinire l'apparato sanzionatorio.

il paragrafo 1 recita: "La presente Convenzione non si applica ai danni da inquinamento contemplati dalla Convenzione sulla responsabilità civile, a prescindere dal fatto che sia o meno dovuto un indennizzo per tali danni in virtù di detta Convenzione". Il paragrafo 2 è quello che desta qualche dubbio che, essendo finalmente il Governo in Aula, potrà essere fugato. In esso si dice: «Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3, le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie e alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un servizio pubblico commerciale», cosa che non appare, almeno scritta in questi termini, nella versione

Si dice: «*only on Government non-commercial service*». Un conto è un servizio governativo non commerciale, un conto un servizio pubblico che offre il Governo. Non si riesce a capire perché siano state modificate queste queste parole. Non dico che ci sia dietro un disegno, un piano o la volontà di non assumersi le responsabilità al centro di questa Convenzione, visto e considerato che già la Camera dei deputati l'ha votata favorevolmente, però, per fugare ogni tipo di dubbio,

in sede di esame del disegno di legge n. 1811 relativo all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, ricordando il preambolo della Convenzione stessa, in particolare il riconoscimento dell'importanza di definire una responsabilità precisa per tutte le forme di inquinamento da idrocarburi e di prevedere nel contempo un'adeguata limitazione di tale livello di responsabilità, nonché la necessità di adottare misure complementari per garantire il pagamento di un indennizzo adeguato, rapido ed effettivo dei danni causati dall'inquinamento derivante da fughe o scarichi combustibili delle navi; considerato che l'articolo 4 della Convenzione elenca le esclusioni dalla responsabilità civile per i danni e che al paragrafo 2 le disposizioni della Convenzione non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente a un servizio pubblico commerciale; considerato il ruolo fondamentale svolto dal naviglio militare nel sostegno a emergenze umanitarie e cataclismi naturali, impegna il Governo: a stipulare comunque contratti assicurativi volti a coprire eventuali danni dovuti all'inquinamento da combustibile delle navi anche per dette situazioni particolari».

per portare aiuti e soccorsi a popolazioni che hanno subìto cataclismi - è partita qualche giorno fa una portaerei italiana per Haiti - oppure nei casi in cui vi siano

L'interpretazione che ci è parso di poter fornire è che dovessero intendersi prestazioni in qualche modo riconducibili ad interventi di protezione civile.

le ragioni. Il senatore Perduca ha chiaramente individuato, nell'ordine del giorno G101, le attività non commerciali del naviglio militare. nasce dal fatto che gli impegni vanno assunti quando è possibile farlo; faccio presente al senatore Perduca che, nel caso di specie, è assolutamente impossibile fare una previsione di spesa degli oneri che maturerebbero qualora

il Governo non ha dato risposte certe in sede di dibattito in Commissione. Abbiamo tutti fatto uno sforzo, a partire da chi ha avuto per primo questa curiosità, cioè chi parla, nel tentativo di interpretare cosa si volesse

Signor Presidente, onorevoli senatori, la tutela del territorio e del mare è argomento attualissimo, non solo per le cronache che abbiamo letto su tutti i giornali, ma anche e soprattutto perché,

di inquinamento. L'inquinamento marino è una delle questioni ambientali più urgenti del nostro tempo e mi riferisco all'introduzione diretta o indiretta da parte umana di sostanze o di energia nell'ambiente marino che provoca effetti deleteri quali danni alle risorse viventi, rischio per la salute umana, ostacolo alle attività marittime compresa la pesca, deterioramento della qualità dell'acqua e riduzione delle attrattive ambientali e turistiche. La tutela dell'ambiente rappresenta una delle sfide globali che richiedono oggi il nostro impegno anche in Parlamento. Anche se il trasporto marino non è tra i fattori più alti d'inquinamento, tuttavia, se sommato all'inquinamento da attività illegali e agli incidenti, determina un quadro preoccupante per l'Italia e per l'intera comunità internazionale. L'Italia arriva con un certo ritardo all'appuntamento con l'adesione a questo protocollo, ma credo che sia importante farlo in maniera convinta e immediata. L'adesione alla Convenzione comporterà anche un impegno nella cooperazione internazionale a livello tecnico, nella prevenzione, nelle operazioni di recupero e salvataggio e nel perseguire eventuali responsabilità civili e penali. L'adesione italiana a questa Convenzione rappresenta, inoltre, un invito a fare meglio e fare di più anche nella lotta a tutte le altre forme di inquinamento del mare, oltre che il contrasto alle attività illegali che contribuiscono ulteriormente all'inquinamento ambientale. Voteremo, dunque, a favore di questo provvedimento che, oltre ad essere un importante strumento legislativo nella lotta all'inquinamento e oltre a tutelare l'ambiente e il territorio, difende le nostre coste e le attività turistiche, unico vero bene economico non delocalizzabile, per cui abbiamo il dovere di fare sempre di più.

Regolare, prevenire e sanzionare i danni che derivano dall'inquinamento prodotto dal combustibile delle navi è fondamentale per un Paese come l'Italia che, data la sua conformazione geografica, risente in special modo del problema del deterioramento dell'ambiente marino. Oltretutto la Convenzione è già stata ratificata da 44 Stati membri e quindi può divenire fin da subito operativa. L'inquinamento marino, come anche i recenti casi di cronaca hanno dimostrato, rappresenta un problema cruciale dei nostri anni, non solo per gli ambientalisti, ma anche per tutti i cittadini, poiché compromettere mari e coste tramite l'emissione diretta o indiretta, da parte umana, di sostanze o di energia nell'ambiente genera effetti che toccano molti campi della vita sociale ed economica. Innanzitutto i danni alle risorse viventi che popolano il mare, quindi un forte rischio per la salute dell'uomo, ma anche, da punto di vista economico, un impedimento alle attività marittime in genere, che siano la pesca, la coltura marina o il turismo. Ecco perché urge la necessità di adottare ogni strumento per tutelare il prezioso patrimonio di cui il nostro Paese è dotato e su cui prospera. Associandomi alle considerazioni mosse dai colleghi dell'Italia dei Valori alla Camera, sottolineo come sia importante non solo che si fissino norme severe, ma anche che queste norme vengano concretamente applicate. E non solo tramite le sanzioni dopo che i disastri ambientali si sono verificati, ma anche e soprattutto tramite una costante e puntuale attività di controllo preventivo; ciò, in riferimento al fenomeno dello sversamento abusivo dalle navi, le quali, al fine di non dover sopportare i costi che i lavaggi impongono se eseguiti a norma di legge nei porti, utilizzano come discarica proprio i mari. Concordo, infine, con la questione posta dal collega Perduca, circa l'esenzione dalla Convenzione di navi militari o altre navi che uno Stato può adibire a servizio pubblico non commerciale. Credo che su una materia tanto delicata come quella del danno ambientale da inquinamento, lasciare tale eccezione, tale impregiudicatezza per le attività statali, sia una leggerezza che dovrebbe essere evitata.

Signor Presidente, evidentemente su questo provvedimento ci sarà un voto favorevole dal parte del Gruppo della Lega Nord Padania. Non voglio comunque essere ripetitivo, considerata l'esposizione

ogni Stato contraente deve accertarsi che ogni nave che entri nei propri porti o che da essi parta sia in possesso dell'assicurazione o comunque di una garanzia. ricordato che milioni di abitanti vivono lungo i 46.000 chilometri di costa del Mediterraneo, nel quale ogni anno vengono riversate 120.000 tonnellate di oli minerali, 60.000 tonnellate di detergenti, 100 tonnellate di mercurio, 3.800 tonnellate di piombo, 3.600 tonnellate di fosfati, a cui si aggiungono plastiche e materiali non biodegradabili. Dal punto di vista ambientale, quindi, la situazione è grave e l'inquinamento ne peggiora ulteriormente le sorti, tenendo presente che il Mediterraneo completa il ricambio totale delle sue acque in circa settant'anni. La Convenzione evidentemente non incide solo sul nostro mare, ma per quanto ci riguarda è corretto tenere in considerazione questi dati e riflettere sulla sorte delle nostre acque. La Convenzione è fondamentale perché va a colmare una lacuna nella disciplina internazionale proprio in questo ambito ed è quindi vitale che il nostro Paese aderisca e aderisca con forza. Il controllo, però, deve avvenire non solamente nei tratti di mare vicino alle coste, bensì all'interno del bacino e ciò significa dare priorità in particolare all'accertamento dell'assicurazione. Dobbiamo renderci conto che per un Paese come il nostro, circondato in buona parte dal mare, l'inquinamento marino è un fenomeno da combattere e l'adesione alla Convenzione in esame ha proprio tale finalità. Pertanto la Lega Nord vota, con convinzione, a favore.

Signor Presidente, ringrazio il collega Bettamio per aver accolto la mia richiesta di poter svolgere un breve intervento in dichiarazione di voto su questo importante provvedimento, che naturalmente apre la strada ad una tematica di grandissima delicatezza.

a questa preoccupazione abbiamo il dovere di segnalare che occorre una maggiore attività, sia sul fronte interno che su quello internazionale. Il mare non conosce confini amministrativi le cause di inquinamento che lo affliggono devono riguardare tutti i Paesi rivieraschi. Auspichiamo che l'attività internazionale del nostro Paese, già fortemente improntata ad una nuova politica mediterranea, possa occuparsi anche dell'aspetto della salute del Mar Mediterraneo, che mi sembra assolutamente prioritario rispetto anche ad altre tematiche pur sensibili e importanti che riguardano tutti i Paesi che vi si affacciano. Il mio Il mio auspicio nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo PdL a questo disegno di legge, quindi, è che si accentui l'attenzione del nostro Governo e di tutti i Governi che fanno parte tanto dell'Unione europea, quanto dell'Unione per il Mediterraneo sulla tematica ambientale riguardante proprio l'equilibrio dell'ecosistema mediterraneo. Per quanto mi riguarda, la 13a Commissione ha già avviato un'indagine sull'argomento, che spero possa contribuire ad una iniziativa che sia di complemento a quella che stiamo oggi esaminando e che veda

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi l'Aula del Senato inizia l'esame del disegno di legge n. 1771 sulle cure palliative e la terapia del dolore, proveniente dalla Camera Affrontiamo così un tema che tocca nel profondo la dignità umana nel momento più difficile dell'esistenza (la sua fine) e nel rapporto drammatico con il dolore fisico. Dalla Camera ci giunge un buon disegno di legge; si tratta di un testo che vede numerosi aspetti positivi. Nell'identificazione del servizio e nella formulazione della sua struttura vediamo una ben precisa concezione del sostegno alla persona malata, che viene collocata all'interno del contesto familiare e delle strutture sociali. L'offerta dei servizi è stata inoltre ancor meglio articolata, anche grazie al lavoro emendativo in Commissione, attraverso due reti distinte: una rete nazionale per le cure palliative e una rete nazionale per la terapia del dolore. La struttura a rete si pone come la migliore risposta alla domanda di servizi sul territorio, perché capace di mobilitare tutte le risorse che compongono un servizio complesso come l'offerta di cure palliative e terapie antalgiche e di ottimizzarne la gestione sul territorio. Questa struttura di erogazione è volta a garantire la continuità assistenziale del malato dall'ospedale al suo domicilio ed è costituita dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle Regioni, dedicati all'erogazione delle cure palliative e al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia. Si creeranno quindi *hospice*, servizi di assistenza domiciliare, *day* *hospice* e centri di assistenza specialistica di terapia del dolore. Un elemento positivo non secondario di questo disegno di legge è poi quello relativo alla comunicazione. Nel testo, infatti, sono previste campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private, nonché delle organizzazioni private senza scopo di lucro. Dunque, non è una comunicazione orientata solo all'informazione, ma anche a rendere consapevole l'opinione pubblica di questa realtà. Infatti, le campagne promuovono e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative, anche pediatriche, e delle terapie antalgiche, al fine di promuovere la cultura della lotta contro il dolore e il superamento del pregiudizio relativo all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento dello stesso, illustrandone il fondamentale contributo alla tutela della dignità della persona umana e al supporto per i malati e per i loro familiari. In Commissione si è lavorato poi sul progetto «Ospedale-Territorio senza dolore» e sull'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno di tutte le cartelle cliniche. Abbiamo approfondito gli aspetti dell'organizzazione dell'Osservatorio nazionale del rapporto con quelli regionali e, soprattutto, si è lavorato con efficacia per semplificare - e lo sottolineo - le procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore. dolore. La semplificazione è certamente un punto fondamentale di questa legge, che permetterà di evitare ai pazienti e ai loro familiari, in un momento così difficile della vita, quell'*iter* burocratico, complesso e drammatico tra centri specialistici, medici di base e farmacie, e porterà anche facilitazioni e garanzie per tutti quegli operatori che in questa procedura terapeutica sono coinvolti, siano essi medici o farmacisti. Quindi, alla ricetta in triplice copia a ricalco, assai complicata nella formulazione e prescrizione, viene sostituita la semplice ricetta del Sistema sanitario nazionale a disposizione di tutti gli operatori. Onorevoli colleghi, permettetemi...

Onorevoli colleghi, permettetemi in conclusione di ringraziare i tecnici del Ministero della salute, del Dipartimento per le politiche antidroga

e tutti i componenti della Commissione di ogni schieramento politico per il clima di fattiva collaborazione durante i lavori di approfondimento del testo. Penso che coloro che hanno partecipato a questi lavori, i membri della Commissione, i tecnici e tutti i colleghi che parteciperanno a questo dibattito, che analizzeranno e approfondiranno questo testo, non solo stiano contribuendo a realizzare una buona legge, ma stiano dando un serio aiuto alla persona malata, alla famiglia in difficoltà e alla dignità dell'uomo che soffre, nel momento più difficile della sua esistenza.

colleghi, con l'approvazione di questa legge e successivamente con la sua applicazione (che noi ci auguriamo sia ampia ed estesa su tutto il territorio nazionale) il nostro Paese compie un passo in avanti molto importante sul terreno dei diritti umani e sociali. Lei, prima, giustamente, ci ha richiamato all'attenzione su questo tema così importante e sul fatto che oggi non stiamo discutendo un provvedimento qualunque, qualunque, ma una legge che incide sulla vita delle persone e sul loro diritto di esseri umani. Sconfiggere il dolore quando questo rischia di rubare la dignità, ricevere aiuto e sostegno nella fase finale della vita, non essere abbandonati, avere accanto a sé la famiglia nel momento della morte: sono diritti umani e sociali, sono bisogni che purtroppo la nostra società spesso non soddisfa e che invece una società moderna, attenta alle persone, dovrebbe soddisfare. purtroppo, in un'epoca in cui tutto deve essere fatto in tempo reale e ciò porta a dedicare molto meno tempo alla cura e agli affetti; per questo spesso è molto difficile per la famiglia del malato terminale reggere al bisogno di cura, di umanità e di dedizione che la fase che precede la morte richiede. Ed è per questo che anche la famiglia deve essere sostenuta nel momento in cui si trova ad assistere il malato terminale, che un numero sempre maggiore di persone muoiano sole e abbandonate in un'anonima corsia di ospedale, senza un'adeguata assistenza, non dico medica, perché questa non viene mai a mancare, ma anche psicologica e di tipo culturale. Il nostro Paese sconta un forte ritardo sia per quanto riguarda la cura del dolore e l'importanza di fare questo tipo di assistenza, sia per quello che riguarda le cure e il sostegno nel fine vita. Solo in questi ultimi anni sono state poste le basi per una buona assistenza ai malati in fase terminale e a quelli con malattie croniche degenerative e tumorali portatrici di un dolore severo,

(e poi ancora nel 1999 e nel 2000) attraverso una serie di raccomandazioni ha chiesto agli Stati membri di operare per il rispetto e la protezione della dignità della persona nella fase terminale di una grave malattia o nel fine vita. Ha chiesto di adottare delle misure legislative o anche di altro genere per sviluppare una rete nazionale diffusa e omogenea di cure palliative, nonché di promuovere i rapporti internazionali al fine di creare una rete tra organizzazioni, istituti di ricerca e altri soggetti operanti nel settore delle cure palliative. Quindi, l'Europa ci ha richiamato da oltre un decennio ad un compito che noi stiamo svolgendo solamente oggi, ci auguriamo, in modo positivo.

spesso in carenza di risorse. Questo lavoro ha consentito al nostro sistema sanitario di porre le basi per lo sviluppo di una buona assistenza ai malati terminali. Vorrei ringraziare anche le tante associazioni di volontariato, spesso prive di risorse e operanti nell'assoluta indifferenza, che hanno svolto un'assistenza ai malati terminali, spesso anche a domicilio quando questi malati non potevano accedere alle cure ospedaliere, con grande spirito di sacrificio e grande capacità umana di sostenere le persone nella fase che precede la morte. una legge, quindi, che deve dare un riconoscimento e una struttura organizzativa diffusa ed integrata sul territorio alle cure palliative e alla cura del dolore.

Ciò che ci stava più a cuore è che fosse riconosciuta l'importanza di costituire due reti, una riferita alle cure palliative e l'altra alla cura del dolore, che fosse riconosciuta l'importanza decisiva del lavoro svolto dai medici palliativisti che sono stati innovatori e costruttori, insieme ad altre figure mediche ed infermieristiche, qualificata seppure ancora insufficiente, presente sul nostro territorio. Un'altra questione per noi importante era relativa alla semplificazione nell'accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore. Purtroppo solo in questi ultimi anni, grazie a provvedimenti dei Ministri della salute, tra cui ricordo il professor Veronesi, si è operata una semplificazione per consentire ai medici di prescrivere medicinali per il controllo del dolore severo. Prima, le difficoltà di accedere ai ricettari preposti era tale che scoraggiava il medico alla prescrizione. Certo non era solo questo il problema, ma anche una cultura che sottovalutava il dolore e lo accettava come una fatalità, che lo vedeva come un dato ineluttabile nella vita delle persone,

Avremmo voluto una maggiore attenzione nell'assicurare l'inserimento nei servizi di cure palliative dei medici che finora sono stati la spina dorsale di questi servizi, insieme al personale

connessa dei servizi preposti, in questo caso alla distribuzione dei medicinali o alla loro prescrizione. Avremmo voluto quindi più coraggio, ma credo che la soluzione trovata sia un grande passo in avanti. Queste sono le questioni più importanti, signor Presidente, e le valutazioni più significative che abbiamo fatto. Certo, sarà molto utile - io credo - dare spazio anche ad una nuova cultura, a quella dell'ospedale senza dolore.

e spesso abbiamo chiesto che ci fosse attenzione a questo tipo di dolore, che ci fossero servizi e attività preposte a ciò, ma il risultato è stato fino ad oggi estremamente limitato rispetto all'impegno che l'Aula ha posto su tali questioni. Riteniamo quindi importante svolgere un'ulteriore azione di sollecitazione allo sviluppo di una cultura dell'ospedale senza dolore e l'informazione, che è una parte importante della legge, potrà - credo - aiutare a sviluppare questo tipo di cultura anche tra i cittadini, al fine di non aver timore di chiedere di non soffrire,

ci appassioniamo alla modifica persino di una virgola, ma poi non siamo in grado di realizzare un controllo su quanto avviene a valle dell'approvazione delle leggi. In tale caso, essendo questo un argomento importante e decisivo per la qualità della vita, per l'umanità, per la crescita di una cultura della cura e dell'affettività tra le persone, dovremo essere molto attenti

con un'architettura internazionale che da 49 anni regolamenta la presenza nel mondo, nel tentativo di controllarla, delle piante, e dei loro derivati, che possono produrre sostanze sicuramente tossiche (le cosiddette droghe e le sostanze stupefacenti) ma, allo stesso tempo, medicine e per l'appunto tutti i derivati che in parte sono già utilizzati nella cura del dolore. Nel 1961 la comunità internazionale adottava la prima Convenzione delle Nazioni Unite per il controllo delle sostanze psicotrope, nella quale dove però in maniera arbitraria si elaboravano quattro tabelle che mettevano sotto strettissimo controllo tanto le piante quanto i derivati. Ne deriva quindi che la canapa indiana, il papavero e la foglia di coca sono trattate alla stregua dei loro derivati, sia che si tratti di derivati fortemente tossici sia che si tratti di derivati da cui si possono produrre anche delle medicine. medicine. Tale architettura, che poi con gli anni è stata ulteriormente rafforzata con altre due Convenzioni, nel 1971 e nel 1988, che hanno ulteriormente ristretto l'ambito in questione, in questione, è stata poi declinata a livello nazionale con l'incorporazione di queste norme nei vari Stati che hanno ratificato i documenti. L'Italia - ahinoi! - alla fine degli anni Ottanta

Le Nazioni Unite, dopo aver adottato questi tre documenti, hanno creato anche un'agenzia specifica, che ha sede Vienna e che l'Italia negli ultimi 25 anni ha sempre diretto con varie personalità (oggi c'è l'economista Enrico Maria Costa), che cerca, da una parte, di farsi garante delle Convenzioni e, dall'altra, insieme alla Giunta internazionale per le sostanze stupefacenti, di regolamentare possibile all'interno delle convenzioni, e cioè una produzione sia delle piante che delle sostanze raffinate per fini medici e scientifici, tra i quali rientrano chiaramente sostanze come la morfina, la codeina ed i derivati della canapa indiana e della foglia di coca.

Al momento in cui si decise di regolamentare la presenza di queste piante nel mondo si fece la fotografia e si disse che l'80 per cento della produzione mondiale di questa pianta doveva rimanere possibile in questi due Stati e che le quote eccedenti potevano essere distribuite in giro per il mondo. Si fecero avanti l'Australia (forse non tutti sanno che l'isola della Tasmania è il più grande produttore di papavero che poi viene utilizzato per l'oppio), ma anche l'Europa:

far rientrare all'interno dell'architettura legale nata con la Convenzione del 1961. Quindi stime, molto spesso stime di stime, perché sappiamo che nel 1961 - ma anche oggi - un terzo dei Paesi facenti parte delle Nazioni Unite non possono essere considerati,

dato alle Nazioni Unite, e lo stesso dicasi per tutta l'Africa subsahariana. Allo stesso tempo, credo che sia impossibile ritenere che in quei Paesi non esista il dolore o, addirittura, che non esistano quelle poche sostanze che possono essere utilizzate per la cura dello stesso.

stabilisce le quantità che legalmente possono essere prodotte nel mondo, sulla base dei dati che vengono forniti dagli Stati a Vienna.

simili, salvo delle piccole eccedenze che possono essere stoccate in luoghi che sono molto più vicini a delle basi militari che non a dei veri e propri magazzini: stiamo parlando infatti di sostanze che, se deviate in alcuni contesti e ulteriormente raffinate, possono sicuramente diventare sostanze tossiche anche letali, come per esempio l'eroina.

rendere molto più facile la prescrizione di analgesici derivanti dalle sostanze catalogate nelle tabelle della Convenzione ONU del 1961 sulle sostanze psicotrope, è chiaro che la domanda reale

tutto questo debba essere tenuto in conto, non perché siano dei ragionamenti astrusi, ma perché se un domani l'Italia dal 150° posto - qual era l'ultima volta che ho controllato le classifiche relative

di oppiacei, ma anche di derivati dalla canapa e un domani, chissà, anche di derivati dalla foglia di coca, perché questo non è che un primo passo verso una direzione che può rendere sempre più possibili e diffuse queste sostanze nel nostro Paese.

al quadrato" o "x al cubo", non so se l'Italia legalmente riuscirebbe facilmente ad approvvigionarsi di queste sostanze senza mettere mano alla legge nazionale che le consente di comprare più morfina rispetto a quella prevista per l'anno in corso

*boom* di domanda di sostanze oppiacee. Tutto questo dev'essere preso in considerazione e mai però è emerso nel dibattito che è stato fatto in Commissione in maniera un po' affrettata, visto e considerato che ieri è stato concluso alle ore 15,30 e abbiamo avuto cinque ore scarse per preparare i documenti. È un peccato che non sia in Aula il sottosegretario Mantica, perché questo ha a che fare con la nostra presenza all'interno dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine di Vienna e avrà a che fare magari, se l'Italia riterrà di prendere in considerazione questi nostri suggerimenti contenutinelle cinque pagine di ordine del giorno che ho preparato insieme alla senatrice Poretti, con la 53a sessione della Commissione droghe di Vienna che si terrà a metà marzo. È lì che la questione va sollevata

per tanti motivi, e non perché si vogliano legalizzare le droghe (anche se noi, antiproibizionisti radicali, le vogliamo legalizzare per regolamentarle: ma questo è un altro tipo di problema), ma perché si ritiene che la quantità di piante e loro derivati prodotti per uso medico e scientifico debba essere aumentata. In Italia, per consentire questa presenza legale e regolamentata, abbiamo cambiato nei mesi di gennaio e febbraio la nostra legge e, quindi, da domani l'Italia vuole avere una quantità di sostanze per la cura del dolore pari a quella degli Stati Uniti. Questo va a sconvolgere gli equilibri a livello internazionale. Non è che noi abbiamo una risposta dal punto di vista

Posto appunto che però va sollevato il problema della modifica di questo meccanismo che bilancia le quote legali di produzione, di acquisto e distribuzione dei derivati delle sostanze contenute nelle convenzioni delle Nazioni Unite, occorre andare a trovare nel mondo chi possa fornirle qualora tutti gli altri 26 Stati dell'Unione europea dovessero adottare una legislazione simile alla nostra. In effetti, i Paesi nordici già l'hanno ora, è più facile essere curati con morfina e codeina, ad esempio. In alcuni Stati, inoltre, si iniziano ad utilizzare i derivati della canapa indiana (e noi abbiamo presentato anche degli emendamenti in questo senso).

perché fanno del bene e addirittura cancellano il dolore. Noi riteniamo, in maniera non provocatoria, ma per il governo di un fenomeno che ha, se non altro, due aspetti, quello delle cure palliative e quello geopolitico e geostrategico, proprio in vista della Conferenza che si terrà a Londra il 28 gennaio sull'Afghanistan, di concerto con gli altri *partner* europei, debba assumersi la responsabilità di proporre la possibilità di trasferire nel mercato legale tutto l'oppio che viene prodotto in Afghanistan; altrimenti si è certi (checché ne dicano gli ex zar antidroga come l'europarlamentare dell'Italia dei Valori Pino Arlacchi, qualcuno che è stato sospeso dalle Nazioni Unite per la sua mala condotta, o anche l'attuale direttore dell'ufficio di Vienna, dottor Costa, che ritiene che la situazione sia sotto controllo) che questo altro oppio verrà trasferito nei laboratori che sono presenti in Afghanistan e nei Paesi limitrofi, trasformato in eroina per essere poi sicuramente venduto nelle *ex* Repubbliche sovietiche e in Europa. Si compri, quindi, si stocchi e si elabori quel derivato del papavero in morfina e codeina e tutti gli altri analgesici oppiacei.

di sei miliardi di persone, neanche un decimo ha accesso facile a questo tipo di cure;

in virtù del nostro tradizionale impegno nei Paesi poveri, specialmente nel settore della sanità, è chiaro che il sistema non regge più.

l'Italia, che promette alle Nazioni Unite di sostenere alcune iniziative ma non sempre mantiene la parola data, la parola data, dovrebbe attivarsi, a parte l'invio delle portaerei, anche con contributi alle agenzie delle Nazioni Unite che si occupano

per la produzione di analgesici; a perseguire politiche che, tenendo conto del contesto nazionale afgano, non avviino l'estirpazione forzata delle colture per non contribuire a creare ulteriori situazioni di conflitto con la popolazione civile, in particolare con le migliaia di contadini che lavorano le migliaia di contadini che lavorano nel settore della produzione di papavero. a iscrivere all'ordine del giorno della 53esima sessione della Commissione Onu sulle Droghe dell'8-12 marzo prossimi la necessità di rivedere in sede multilaterale il meccanismo che alloca le quote di produzione legale del papavero per oppiacei ipotizzando l'inclusione dell'Afghanistan tra i paesi che oggi coprono la cosiddetta domanda legale internazionale.

offro osservazioni aggiuntive rispetto a quelle espresse dalla senatrice Bassoli, che condivido profondamente. Il disegno di legge in esame è importante

serve anche per quei pazienti, come per esempio i pazienti diabetici, affetti da gravi patologie neurologiche: quindi, riguarda un'ampia gamma di persone.

e le loro famiglie che vivono una condizione di dolore e di fragilità. Affrontare il tema delle cure palliative vuol dire quindi parlare del dolore, della dignità che esso deve avere; vuol dire parlare di speranza, di solidarietà, di famiglia, di sostenibilità, di universalità e di uguaglianza. In fondo, il dolore, se lasciato a se stesso, significa abbandono, significa solitudine e può degenerare anche in disperazione, mentre se è accompagnato e intriso di quei valori a cui facevo riferimento prima (speranza, solidarietà, sostenibilità, universalità e uguaglianza) uguaglianza) il dolore diventa un accompagnamento, una condivisione, una responsabilizzazione da parte della società. Il disegno di legge in esame è questo: la società si fa carico delle persone che vivono una condizione di dolore. Il dolore è difficile da comprendere, perché significa accettare il concetto di limite della persona umana.

e la Camera dei deputati ha dimostrato che sono diverse, perché infatti questo disegno di legge alla Camera è stato approvato all'unanimità, mentre il disegno di legge sul testamento biologico ha avuto dei voti diversi qui in Senato (adesso lo stanno affrontando

cosa vogliamo dire alla società dal punto di vista culturale con questo provvedimento, che speriamo diventi il più in fretta possibile legge. Sostanzialmente vogliamo dire che lo Stato, le istituzioni pubbliche, e quindi la fiscalità generale, si fanno carico delle persone che vivono una condizione di dolore, di dolore, nella maggior parte dei casi solo nella fase terminale della vita (in altri casi, invece, il dolore accompagna la loro vita). vita). Il farsi carico significa che la fiscalità generale mette a disposizione delle risorse affinché queste persone possano vedere alleviato il loro dolore. possano vedere alleviato il loro dolore. Accanto a questo, il disegno di legge offre altre scelte, si fa carico di una rete di servizi; infatti, mette a disposizione delle risorse della fiscalità generale per realizzare gli *hospice* sul nostro territorio, ma individua anche le cure domiciliari come un momento importante per andare incontro alle persone che vivono una condizione di dolore. Quindi, una rete di servizi:

Paese. Al Nord, pur essendo in presenza di una carenza, in alcuni casi, di strutture, riusciamo però a soddisfare mediamente al bisogno di cittadini che vivono una condizione di dolore e che sono nella fase terminale della vita attraverso gli *hospice.* Spesso invece in alcune Regioni del Sud i cittadini non sanno neppure dell'esistenza degli *hospice* - il che è gravissimo non conoscono neppure il concetto di cura e di assistenza domiciliare, perché non viene garantito nulla a loro: questo è altrettanto grave

scriva che si è sentito abbandonato nel momento del dolore. Purtroppo invece molti l'hanno scritto, perché si sono sentiti abbandonati.

prevede la somministrazione delle sostanze stupefacenti come sostanze per alleviare il dolore.

non dava la possibilità di usare in modo improprio queste sostanze, dava la possibilità di effettuare tutti quei controlli che, dal punto di vista medico e paramedico, devono essere operati su queste sostanze.

e che hanno bisogno di vedere alleviata la propria sofferenza. Io sono contrarissima all'uso improprio delle sostanze stupefacenti; il mio pensiero diverge radicalmente dal discorso che ha fatto prima

eccessivamente e di complicare per il cittadino paziente l'uso di tali sostanze. Mi rivolgo a tutti i colleghi che vogliono arrivare all'approvazione di una buona legge.

anche questa legge, fra qualche anno, sia ricordata come una buona legge. Ciò vuol dire che i cittadini e le loro famiglie avranno visto uno Stato che avrà dato risposta ai loro bisogni, senza equivoci, senza se e senza ma, senza burocrazie e senza allargamenti impropri. È a questo, credo, che tutti noi vogliamo arrivare. arrivare. Siccome le cure palliative e la terapia del dolore vanno incontro ad una condizione che per il cittadino si ripete,

Ulisse. Vi ricordate la tela di Penelope? Questa donna faceva e disfaceva la tela, perché aspettava il suo Ulisse. Quando Ulisse arrivò

non è risolutivo del suo problema, è solo qualcosa che allevia, che dà una dignità a quel dolore e a quella persona. Noi come Stato dobbiamo essere Argo, dobbiamo mutuare l'esperienza di Argo, dobbiamo continuamente accorgerci che quella persona ha bisogno di noi.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi e colleghe, ogni paziente inguaribile è comunque curabile.

Le cure palliative sono destinate a soddisfare i bisogni del malato e della sua famiglia, non tralasciando nulla di ciò che provoca dolore fisico, psichico e spirituale. Ciò significa prevenire e contenere i sintomi tipici delle malattie irreversibili, ma anche garantire il miglior supporto psicologico, spirituale e sociale alla persona malata e alla sua famiglia. Proprio per questo principio, ogni paziente inguaribile è curabile. Nelle cure palliative l'attenzione è rivolta innanzitutto alla persona, poi alla malattia. Con le cure palliative non si affretta la morte, né la si ritarda, ma si tutela la qualità della vita del paziente e dei suoi familiari. La fine della vita è considerata certamente un processo naturale, ma si trattano con attenzione sia il dolore, sia gli altri sintomi disturbanti. Nelle cure palliative tutti gli interventi devono essere di natura multidisciplinare e gli aspetti psicologici e spirituali rientrano nel piano di cura della persona malata; offrire sistemi di sostegno per rendere dignitosa e attiva la vita del paziente, supportando la famiglia nel corso della malattia. Il tema delle cure palliative e della terapia del dolore è stato caratterizzato da un cammino lungo negli anni, che ha interessato il dibattito emerso nel corso delle più recenti legislature.

sia stato arricchito dal contributo apportato dalla Commissione sanità, della quale faccio parte. L'attuale Governo ha fortemente appoggiato questo disegno di legge, passando dalle parole ai fatti. Se, come ha detto la senatrice Bassoli, il ministro Veronesi è stato tra i primi a mettere sotto i riflettori questo importantissimo aspetto, fino a pochi anni fa trascurato, è stato questo Governo a passare ad una fase

Il Governo ha oltretutto promosso la realizzazione di reti nazionali per la terapia del dolore e le cure palliative. Queste reti nazionali sono volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze individuali. È fondamentale correggere - com'è già stato ricordato - le enormi differenze tra Regione e Regione e tra i vari distretti di una stessa Regione. Le figure professionali (medici, paramedici, assistenti sociali e psicologi) disponibili nelle Regioni e nelle Province autonome e dedicate all'erogazione delle cure palliative e al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alla fase terminale della malattia stessa, devono garantire un'univoca preparazione professionale e culturale, perché ad oggi, in Italia, non esistono tali specializzazioni a proposito di questo delicatissimo fronte. Viene segnalata anche l'importanza che queste cure hanno per i piccoli pazienti in età pediatrica: è molto importante coinvolgere nella formazione la figura del pediatra. Il Ministero della salute ha identificato quattro Regioni pilota (Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Sicilia) come modelli di rete per la formazione della terapia del dolore e una Regione pilota (Piemonte) per la formazione mediante *master* universitari per le cure palliative. L'università di Torino infatti ha attivato, fin dal 1998, corsi di perfezionamento in cure palliative, per arrivare attualmente ad un quarto*master* biennale di formazione, di secondo livello, aperto soltanto ai medici specialisti. L'obiettivo generale dei *master* in medicina palliativa è quello di formare figure professionali idonee ad operare nell'ambiente della palliativa sia da un punto di vista generalistico che specialistico, ponendo attenzione sia alle patologie oncologiche che ad altre (tipo quelle cardiologiche e neurologiche), facendo una preparazione teorico-pratica, consentendo l'acquisizione di strumenti conoscitivi e operativi idonei agli sbocchi occupazionali che si stanno delineando a livello regionale e nazionale per le varie strutture post-acuzie e *hospice*. Credo che le figure professionali che avranno frequentato i *master* formativi dovrebbero avere la possibilità di raggiungere l'abilitazione con un esame di idoneità giudicato da una commissione nazionale. Tra le proposte emerse nel corso del dibattito, come quella relativa alla presenza degli anestesisti negli *hospice*, c'è da sottolineare come meriti un adeguato approfondimento l'analisi del profilo di sicurezza dei farmaci antidolorifici, con particolare riferimento a quelli di derivazione oppiacea, affinché non si arrivi a sottovalutarne i potenziali rischi in assenza di un sistema sistema attento di monitoraggio. Molto importante è la campagna informativa prevista dal disegno di legge, come è fondamentale e innovativa la segnalazione in cartella clinica e la creazione di un osservatorio per monitorare la rete sul territorio. Le strutture dedicate alle cure palliative, anche interne agli ospedali, devono essere gestite da un gruppo specializzato di operatori professionali, volontari compresi, che hanno funzione di integrazione e di supporto.

Gli *hospice* devono essere quindi un ricovero temporaneo o permanente per le persone malate che non possono essere più assistite con un programma di assistenza domiciliare specialistica o per le quali il ricovero ospedaliero non è più sufficiente. Ricordiamo la visita del Santo Padre ad un *hospice* romano a considerazione dell'importanza del fattore dolore nella vita umana. Il pensiero del legislatore dovrebbe essere sempre volto al benessere e alla salute dei cittadini, soprattutto di quelli che, come in questo caso, già soffrono a causa di uno stato di salute debilitato e vacillante, affinché proprio in questa fase dolorosa e difficile non si sentano abbandonati a sé stessi, bensì al contrario sostenuti, accompagnati e incoraggiati, e questo pensiero è stato tradotto in realtà dall'intervento del nostro Governo, presente oggi nella persona del ministro Fazio, che ringrazio.

ritengo avesse ottime possibilità per vedere una corrispondente situazione di unanimità anche al Senato, ha però visto un *iter* che, secondo me, non ci fa onore come Parlamento. Questo testo è stato assegnato alla Commissione sanità alla fine di settembre; tale Commissione si è evidentemente occupata, prevalentemente e ossessivamente, di un'unica da settembre a dicembre, che è stata un'indagine conoscitiva sulla pillola abortiva RU-486. Questo disegno di legge è stato pertanto accantonato; a dicembre l'abbiamo ripreso, fissato nottetempo il termine per gli emendamenti in Commissione, votati subito alla ripresa dei lavori, e ieri, l'ultimo atto - a mio avviso - di spregio alle istituzioni è stato che questo testo è uscito dalla Commissione alle ore 15,30 e alle ore 20 veniva fissato il termine per gli emendamenti per l'Aula. Io, che ho seguito i lavori in Commissione, ho visto in due giorni il testo cambiare radicalmente - non sempre in negativo, anche in positivo, ma comunque cambiare - in tutti gli articoli,

una lettera, di un testo unico sugli stupefacenti che a sua volta nel corso degli anni è stato modificato crea una legge di difficile interpretazione. Allora, io l'ho capita così

con qualsiasi tipo di ricettario (quello speciale per gli stupefacenti, quello rosso del Servizio sanitario nazionale e perfino quello bianco) potevano prescrivere perfino la morfina per via endovena, anche a domicilio.

era il testo della Camera. Quello che è uscito ieri pomeriggio alle ore 15,30 sinceramente non l'ho ancora ben capito, anche perché non ho avuto il tempo di rifare tutto quel giro di palliativisti e di esperti del settore che ne diano una corretta interpretazione. si sia arrivati alla conclusione che la ricetta, oltre a quella speciale per stupefacenti, è anche quella rossa, cioè quella in carico al Servizio sanitario nazionale.

se non credo che un parlamentare si debba affidare e fidare di un Ministro, ma non perché io sono dell'opposizione e lui è della maggioranza, ma solo perché non credo sia questo il compito del legislatore, né tanto meno quello di fare leggi interpretabili; infatti, se il testo già è interpretabile qui,

È solo un problema culturale? Non credo che gli italiani provino piacere a soffrire, non soltanto nella fase terminale della loro vita, cosa che comporta terapie palliative,

se si vieta la sostanza, ma non l'uso della sostanza, nei fatti si mette lo stigma alla sostanza e se ne impedisce poi la diffusione, la promozione e quant'altro.

proibite, ma alle quali viene riconosciuta un'attività farmacologica - debba sentire il Consiglio superiore della sanità - ed

e a sottolineare io stessa quanto spesso esse si possano intersecare. Secondo studi scientifici, riviste scientifiche riconosciute dalla comunità internazionale e oltre 17.000 studi, queste terapie aiutano per elencarvi possono aversi delle ricadute positive attraverso i principi attivi della *cannabis*. malattie infiammatorie croniche intestinali (morbo di Crohn, colite ulcerosa); tumorali; lesioni midollari; malattie neurodegenerative (morbo di Alzheimer, corea di Huntington, morbo di Parkinson); epilessia; malattie autoimmuni (lupus eritematoso); sindromi ansioso-depressive; patologie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, aterosclerosi); sindromi da astinenza nelle dipendenze da sostanze da abuso (alcool e fumo).

post-traumatico che colpisce frequentemente i militari di ritorno dalle zone calde di guerra e che subiscono traumi per combattimenti ed attentati terroristici. Da qualche anno il Governo israeliano sta utilizzando questi principi per i propri militari,

inserito nella tabella 2. Gli studi stavano a testimoniare che aveva effettivamente una riconosciuta attività farmacologica. Dopodiché siamo in uno stato di limbo, per cui a quel principio è riconosciuta un'attività curativa medica,

sentire il proprio medico, passare attraverso l'ASL, seguendo un *iter* burocratico davvero complicato e alla fine importarlo dall'estero. Questo avviene per terapie che non durano più di due mesi.

In alcuni casi ci sono pazienti fortunati, pochissimi in Italia, che appartengono ad alcune ASL che hanno deciso di rimborsare tale farmaco;

se io lo compro attraverso questa procedura mi costa 600 euro; se io quella stessa pianta la coltivo a casa finisco in carcere per coltivazione illegale di stupefacenti.

Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, vorrei sottolineare con questo mio intervento soprattutto gli aspetti positivi e costruttivi di questo disegno di legge, che aveva come finalità quella di attenuare il dolore e migliorare le terapie dei malati dei malati veri. Finalmente, infatti, arriva al traguardo una legge che reca disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alle terapie del dolore; finalmente, dico, perché si riconosce qui una dignità, ma anche una specificità, a un settore che è sicuramente tra i più importanti nel campo medico e certo tra i più delicati. È un provvedimento importante perché si rivolge a chi non ha più una cura specifica,

importante perché anche il dolore non risolto, il dolore non tumorale, fa spesso perdere la dignità alle persone. Quindi, non è pensabile che il dolore non sia affrontato anche negli ospedali in cui si fa un battaglia particolare contro il dolore come i nostri. È una legge di civiltà, che riconosce le necessità del tempo presente, non è una legge astratta

per ampliare il campo di intervento del nostro sistema sanitario, determinandone un percorso e anche dei paletti in modo preciso. In modo corretto, a mio avviso, si definiscono le professionalità e si identificano due reti separate tra di loro. È sicuramente giusta questa divisione, anche se, come tutte le divisioni fatte in medicina e in sanità,

stia assolvendo sostanzialmente al proprio dovere. C'era la necessità di una legge sulla terapia palliativa e sulla terapia del dolore che ormai era attesa da tempo. Il relatore ha fatto bene a ricordare che il testo che oggi discutiamo in Aula è un testo unificato proveniente da diverse proposte di legge che erano state presentate nel corso degli anni. È, quindi, una legge attesa da tempo dal nostro Paese

ai malati terminali e cronici in fin di vita per rimetterli al centro dei servizi sanitari nei tempi, nei luoghi e nelle modalità di cui loro hanno realmente bisogno insieme alle loro famiglie. Noi, con questo provvedimento di legge, in fondo non concediamo nulla di più di quanto si stia già facendo e di quanto si sia già fatto in molti Paesi europei.

a una lettura più attenta e più profonda, parla soprattutto di dignità e di qualità della vita umana, di assistenza nel rispetto della dignità umana. È questo in fondo quello che ci viene chiesto dall'Europa

ma come assistenza ai bisogni affettivi, psicologici e sociali di tanti malati che si trovano in queste condizioni.

abbiamo infatti 150.000 malati che ogni anno dovrebbero entrare nel programma delle cure palliative. Questo però non è possibile non solo perché mancano i mezzi economici, mancano - da oggi dovremo cominciare a lavorare in questo senso - le strutture, la formazione del personale, la preparazione di personale adeguato che possa rispondere in maniera adeguata a questo bisogno di assistenza. Sempre nel nostro Paese da 50.000 a 80.000 persone l'anno muoiono con dolore. Questo accade non perché non vi siano mezzi terapeutici per far fronte al dolore, ma semplicemente perché non c'è un'adeguata preparazione all'assistenza medica e strutturale della terapia del dolore.

bambini che, anche tramite le strutture che questa legge metterà a disposizione, dovranno aver bisogno dell'assistenza alle terapie terminali (è un dato, comunque, sconvolgente che fa rendere conto a tutta l'Assemblea della delicatezza e della complessità della materia di cui stiamo parlando oggi). C'è un altro dato che mi sconvolge, signor Ministro

a sopperire alla necessità di creare un modello assistenziale nuovo, più complesso, moderno ed adeguato.

in precedenti piani sanitari e dispositivi di legge: il Piano sanitario nazionale 2003-2005 la stessa legge 8 novembre 2000, n. 328, e i successivi decreti attuativi, contenevano importanti indicazioni alle Regioni finalizzate a raggiungere la piena integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale per l'assistenza domiciliare. modo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 (si tratta di nove anni fa) già individuava

motivo è importante ricordare - come è stato fatto autorevolmente da altri colleghi - che il nostro Paese, secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Associazione italiana di oncologia, è agli ultimi posti nell'utilizzo di farmaci oppiacei e oppioidi nel controllo e nella terapia del dolore. Quindi, è un piccolo passo avanti nel consentire una migliore semplificazione della materia, una maggiore accessibilità ai medici nel far uso di farmaci che servono a tenere

prestabiliti annualmente per questo grande e straordinario progetto obiettivo sono ancora insufficienti, anche perché non possiamo lasciare tutto all'autonomia delle Regioni,

ad adempiere ai livelli minimali di assistenza. Su questo il Governo nazionale dovrà vigilare, signor Ministro. Il progetto è di straordinaria portata non solo per solo per la quantità di cittadini interessati, ma soprattutto per la materia che affronta. Noi dell'Italia dei Valori vigileremo sul monitoraggio che il Governo dovrà effettuare sulla rete esistente; vigileremo sulla necessità di informazione che dovrà essere data ai cittadini, che è un altro aspetto qualitativo di questa legge;, sulla formazione che si dovrà dare ai medici impegnati nella materia;

Attenderemo il Governo e il ministro Fazio, alla fine di quest'anno, nella Relazione annuale che il Ministro dovrà portare alle Camere su quanto fatto di fronte ad un argomento di così straordinaria importanza.

e alle terapie del dolore. Come prima diceva la collega Bassoli, il dolore non è legato soltanto ai malati terminali, ma esiste anche il dolore, per esempio, dovuto al parto. Il parto indolore, con l'anestesia peridurale, incontra in Italia ancora molti limiti.

Molte Regioni non garantiscono un servizio nel proprio territorio, violando un diritto acquisito delle donne, ma anche una disposizione legislativa nazionale che prevede l'essenzialità di tale livello assistenziale, visto che l'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione degli ospedali territoriali senza dolore, e la lotta contro il dolore è uno dei punti più qualificanti di questo

e che venga garantita la presenza di personale qualificato, quale il medico anestesista e gli infermieri professionali, affinché il parto indolore anche in Italia sia assicurato, come in tutti gli Stati d'Europa, alle donne che ne fanno richiesta. Questo può essere sicuramente un punto molto più qualificante per il nostro Servizio sanitario nazionale.*(Applausi* Signora Presidente, signor Ministro, gentili colleghe e colleghi, una prova di civiltà ed anche di grande responsabilità ci viene consegnata dalla Camera dei deputati e ci viene oggi confermata dal lavoro svolto nelle aule di Commissione e in questa stessa Aula, che si riappropria della sua funzione: quella del confronto come metodo, come sistema per comprendere, per approfondire, per formare un convincimento. E appare anche straordinariamente importante notare come quest'Aula, che ieri ha registrato anche momenti di tensione sconfinata fuori

garbo e cortesia non formali, ma sostanziali nella modalità di confrontarsi e di sforzarsi nel conseguimento di un risultato. Anche l'intervento del collega Mascitelli sintetizza in modo efficace la capacità

perché in modo condiviso, per alcuni versi anche attraverso un confronto serrato, esso ci permette di consegnare al Paese

criticità che vanno ben oltre gli aspetti più evidenti e più percepiti della efficienza dei servizi sanitari e si estendono a quelli che, talvolta, forse sono meno percepiti, meno avvertiti, ma straordinariamente più importanti perché attengono alla dimensione della dignità della persona. Credo che questo provvedimento consentirà al nostro Paese di risalire in fretta la classifica dei livelli di efficacia e di appropriatezza, sia nell'ambito delle cure palliative sia nell'utilizzo terapeutico delle sostanze destinate a controllare il dolore, dove - ahimè - gravitiamo da tempo nei bassifondi della graduatoria internazionale, a distanza siderale dalle posizioni dei Paesi più avanzati e addirittura dietro molti Paesi in via di sviluppo. Una situazione insostenibile non già e non tanto per l'imbarazzante figura di fronte alla comunità internazionale, quanto per le drammatiche conseguenze pratiche: centinaia di migliaia di pazienti - e fra essi anche tantissimi bambini - vittime di inefficienze. Parliamo dei pazienti oncologici, ma anche di pazienti colpiti da lesioni nervose, da traumi o alle prese con i postumi di un intervento chirurgico, rimasti penalizzati da ingiustificate e gravi criticità nei sistemi assistenziali e condannati a a sopportare sofferenze indicibili, nonostante le moderne conquiste delle scienze farmaceutiche ci consegnino opportunità straordinariamente importanti. In Italia ci sono, soltanto per l'ambito di nostro interesse, 250.000 pazienti in fase terminale; di questi, 150.000 sono pazienti affetti da patologia oncologica. patologia oncologica. Soprattutto in questo campo della sanità l'indice di complessità e la domanda di assistenza crescono con una velocità enorme, alla quale sino ad oggi il legislatore non ha saputo adeguarsi e con esso, quindi, né il sistema normativo, né - scendendo per i rami - il sistema della filiera complessiva che eroga le prestazioni. avviene per un approccio, probabilmente anche di tipo culturale, carente e talvolta inadeguato, come dimostra la rigida quanto incomprensibile regolamentazione delle terapie antalgiche, redatta a partire sin dalla legge n.

criteri di contrasto severo e stringente agli illeciti in materia di stupefacenti, che però sembra abbiano inevitabilmente pregiudicato un accesso agevole alla terapia. Né sono state sufficienti le correzioni che nel corso degli ultimi anni sono state apportate apportate alle norme: penso alle leggi n. 12 del 2001 e n. 49 del 2006, apprezzabili ma ancora non sufficienti, troppo lontane dalle esigenze dei pazienti, dei loro familiari, degli operatori della sanità. Mi riferisco in particolare a medici e farmacisti, guardati fino a ieri come potenziali narcotrafficanti, da mettere in condizione di non nuocere, più che sentinelle di un territorio, protagonisti di quel sistema di sanità che grava in termini attuativi sulle loro responsabilità. Di qui la minuziosa normativa sul ricettario speciale, la copiatura a mano, il bollo sulle tre copie di ogni prescrizione; ancora, la previsione di sanzioni penali assolutamente vessatorie anche per gli errori formali, le limitazioni quantitative e temporali dei dosaggi, gli obblighi di conservazione di una documentazione copiosa ed abbondante. Mille vincoli, mille lacci e lacciuoli a nodi stretti, che non hanno certamente portato il Paese in una posizione di modernità e di dignità. Il risultato è evidente, scontato e inevitabile. Prima che fossero introdotte le parziali semplificazioni cui facevo riferimento, in qualche misura propedeutiche alla rivoluzione positiva che rappresenta questa legge, soltanto due medici italiani su dieci (media che nel Sud del nostro Paese scendeva ulteriormente) si preoccupavano di ritirare presso l'Ordine provinciale di appartenenza oppure presso la ASL, come prevedeva la normativa successiva, gli specifici ricettari per la prescrizione di oppiacei. La stragrande maggioranza dei professionisti, pur di evitare l'astruso e penalmente insidioso percorso ad ostacoli (un riflesso difensivo certamente censurabile, ma che sarebbe ipocrita non ritenere almeno comprensibile), preferiva infatti ripiegare su altre terapie, utilizzando dosi massicce di farmaci non specifici (in particolare gli antinfiammatori), di efficacia incomparabilmente inferiore e, per di più, dagli effetti secondari particolarmente pesanti. C'è voluto tanto, anzi troppo tempo; ma oggi disponiamo di regole che finalmente consentono di uscire da quello che per i malati e per i loro familiari era un vero e proprio girone infernale, affollato di veri e propri condannati al dolore. La legge che oggi ci accingiamo ad approvare rappresenta infatti un deciso passo in avanti del nostro Paese in materia di terapia antalgica, con il positivo effetto collaterale di far registrare il confortante dato politico del lavoro condiviso che maggioranza ed opposizione hanno condotto per arrivare a questo risultato. Nel merito, voglio subito dire che l'impianto di questa legge è convincente sin dall'articolo 1, che pone l'accento sulla necessità di tutelare la dignità e l'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione, promuovendo la qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, e garantendo un adeguato sostegno sanitario, socio‑assistenziale e spirituale della persona malata e della sua famiglia. In coerenza con questo principio fondamentale, il provvedimento introduce norme importanti che semplificano l'accesso ai farmaci per la terapia del dolore. Ma ancora, di particolare rilevanza, sembra opportuno citare l'istituzione e l'organizzazione di due distinte reti, una per le cure palliative e una per la terapia del dolore, facenti capo (anche attraverso le previsioni emendative, alcune delle quali approvate) ad un'unica struttura dipartimentale, per agevolare le necessarie attività di coordinamento che sono disciplinate a livello regionale e nazionale, nel rispetto dell'autonomia regionale. A A quest'ultima non poniamo alcuna limitazione, ma rispetto ad essa è necessario rilanciare sotto il profilo della vigilanza e del controllo, signor Ministro, per evitare che questo Paese continui a declinare modalità non solo differenti, ma addirittura divaricate, con una penalizzazione assolutamente ingiustificata,

attraverso questa legge, che supera i deficit strutturali ed organizzativi, crea condizioni di omogeneità applicativa sul territorio, superando i superando i profondi divari tra Regione e Regione, risolvendo le criticità nei percorsi socio-sanitario-assistenziali e creando un virtuoso collegamento attraverso il cosiddetto sistema delle "tre H" (*home*, *hospice,* *hospital*), con un più convinto e concreto coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Parimenti convincenti e necessari sono gli altri aspetti: la definizione dei requisiti tecnico‑strutturali ed organizzativi delle strutture; la considerazione riservata alla formazione professionale degli operatori sanitari, a partire dai medici (tenuto conto che i i vigenti *curricula* universitari non prevedono specifici insegnamenti); la valorizzazione professionale e la tutela lavorativa degli operatori che hanno conseguito sul campo una specializzazione che oggi non esiste a livello di università

una domanda crescente e ad un bisogno assolutamente prioritario); il rafforzamento del progetto «ospedale e territorio senza dolore».

quanto malinteso sentire, anche a livello di pubblica opinione, in ragione del quale troppo spesso i malati considerano normale la sofferenza fisica, un'ineluttabile tributo da pagare alla malattia, e gli stessi medici parole dell'Organizzazione mondiale della sanità - sembrano poco sensibili al problema. Tutto questo non può e non deve più accadere. Mi piace ricordare le parole rivolte da Madre Teresa di Calcutta ad una moribonda. Riferisce Madre Teresa: «Un giorno incontrai una donna che stava morendo di cancro e, vedendola lottare con questa terribile sofferenza, le dissi: sai, questo non è che il bacio di Gesù, il segno che sei giunta vicino a lui sulla croce e che egli ti può baciare. Ella congiunse le mani e mi rispose: Suor Teresa, la prego, dica a Gesù di smettere di baciarmi». Credo sia l'interpretazione più sublime di quanto sia necessario restituire in modo pieno e concreto

più avvertito senso di gratitudine e di compiacimento per la modalità con la quale si sono svolti i lavori, con l'assistenza del Governo, del ministro Fazio, del sottosegretario Giovanardi,

che hanno dimostrato un livello di partecipazione e di preparazione specifica, consentendo di raggiungere questo obiettivo credo, anche con l'approvazione degli emendamenti che sono stati presentati, consegnerà al nostro Paese una legge necessaria, ma soprattutto completa, sulla cui applicazione certamente poniamo